Colleghi, la seduta è sospesa per dieci minuti.

16.500/2, 16.500/3, 16.500/4, 16.500/5 e 16.500/6, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».

Su questa materia si è già intervenuti con modifiche al codice civile nel 2005, non risolvendo il problema e trattandolo in modo parziale. Ora si torna a trattarlo in questo modo, cercando di percorrere una scorciatoia che certamente allungherà la strada. Il tempo per intervenire sulla materia onestamente c'era, non solo in questa legislatura. Sono 21 anni che la prassi del *trust* si è aperta nel nostro Paese e che gli operatori devono ricorrere all'istituto del *trust* retto dalla normativa di altri Stati che lo hanno normato, perché all'interno del nostro ordinamento non è sostanzialmente possibile applicarlo.

Cinzia Fontana ha ricordato i numerosi rilievi tecnici che su questa materia sono stati fatti dagli stessi Uffici

la previsione contenuta nella delega al Governo di perfezionamento del contratto di fiducia con il versamento intero del denaro: quindi, la trasformazione di fatto del contratto di fiducia in un contratto reale, cui consegue come logica conseguenza che il contratto viene meno se non è perfezionato con le modalità qui previste.

anziché semplificare la vita dei soggetti cui riteniamo di dover fornire un nuovo strumento normativo per far fronte ad esigenze che, in alcuni casi, credetemi, sono anche delicate,

il complesso della materia nella sua sede, nella Commissione, dove già sono i disegni di legge; ci impegniamo a definirla in tempi concordati e certi, di modo che il problema della necessità ed urgenza sia così superato; riportiamo al legislatore il compito del legislatore

sono esaurienti. Vorrei dire soltanto che si ritiene di inserire nella legge comunitaria un istituto che finisce col trascinare nell'ambito del nostro sistema il *trust,* perché il contratto di fiducia altro non è che una forma di *trust* italiano. Su questa materia vi sono discussioni che durano da anni, e già in precedenti occasioni, anche in Aula, disposizioni legislative sono state stralciate per approfondimenti. Che cosa è accaduto? Non abbiamo un obbligo comunitario in materia e tanto meno un obbligo in scadenza. Abbiamo, tra l'altro, una sottrazione della materia alla Commissione giustizia, dove pende il disegno di legge governativo recante la delega al Governo per apportare modifiche al codice civile in materia di disciplina della fiducia, ossia l'Atto Senato n. 2284.

si trasferisce un istituto che ha altre tipologie negli ordinamenti anglosassoni, e gli si danno caratteristiche di contratto, con una serie di incongruità che naturalmente renderanno ancora più difficili le attività degli operatori del settore.

la delega appare in più punti particolarmente generica, specialmente là dove autorizza al coordinamento con le norme tributarie e consente di operare deroghe indeterminate alla disciplina di tutela dei creditori, alla disciplina del contratto a favore di terzo, alla disciplina sulla cessione dei crediti futuri ed alla disciplina degli strumenti finanziari. Indeterminata appare altresì l'autorizzazione a derogare alla disciplina fallimentare, né l'articolo in esame pone sufficienti criteri per la revoca del fiduciario. Parimenti in bianco la delega si configura infine nella parte in cui rimette al Governo la scelta dei casi in cui gli effetti del contratto di fiducia possono derivare dalla sentenza del giudice. Tenendo conto del fatto che la delega comprende anche l'ipotesi in cui il titolare dei beni se ne dichiari fiduciario, e palesemente non può configurarsi come contratto, come infatti generalmente non si configura il *trust,* la disciplina della fiducia si applicherebbe anche qualora gli effetti di questa fossero derivati da testamento, l'introduzione nell'ordinamento di una disciplina del *trust* non ben calibrata potrebbe avere, come effetto della eccessiva discrezionalità lasciata al legislatore delegato, una attenuazione dei principi di trasparenza e di prevenzione dell'elusione, che assolutamente debbono presiedere ad uno strumento utile ma delicato come il Esso comporta infine, come effetto, la separazione del patrimonio e la opponibilità ai terzi, di modo che nessuno può rivalersi sul patrimonio del *trust* vantando diritti verso il il disponente. Occorre quindi che la delega sia sufficientemente puntuale, in modo da non lasciare temere anche possibili utilizzi disinvolti del nuovo istituto in riferimento a grandi patrimoni, compresi quelli che hanno fatto ingresso in Italia, almeno sulla carta, a seguito dello scudo fiscale che ha recentemente concluso i suoi effetti. Signor Presidente, illustrerò brevemente l'ordine del giorno G12.100 a firma mia e del senatore Saia. Con questo ordine del giorno,

tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia di fiducia e *trust*, si è in presenza di una regolamentazione normativa e di prassi abbastanza chiara in materia di imposizione sul reddito, mentre sussistono incertezze in materia di imposizione indiretta, cioè imposte d'atto e di successione e donazione,

In questo senso va il nostro ordine del giorno. Riteniamo che la delega dovrebbe essere rafforzata con il riferimento alla disciplina fiscale da coordinare il nuovo strumento con la disciplina vigente che riguarda le imposte sui redditi, colmare le lacune esistenti

sempre con riferimento alla lettera *r)*, che prevede un coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di *trust* - distinguere i contratti fiduciari riconducibili alla fattispecie del *trust*, che per loro natura dovrebbero costituire uno strumento agile, in uso agli operatori economici, per consentire aperture di credito garantite, spostando il momento impositivo dallo spossessamento al trasferimento del bene al creditore o al terzo, e solo quando questo trasferimento si realizza per effetto della escussione della garanzia. Abbiamo ritenuto quindi di ripresentare questo ordine del giorno e ci auguriamo un ripensamento del Governo e quindi un impegno dello stesso in tal senso.

12.202 e 12.203, mi rimetto al Governo. L'ordine del giorno G12.100

un fenomeno giuridico, già da tempo affermatosi nella prassi, nel nostro ordinamento, tramite l'adozione di moduli normativi che vengono da altri Paesi, tanto da richiedere da molto tempo l'adozione di un'apposita disciplina fiscale. Per questa ragione io penso che la delega sia necessaria.

un impegno sulle indicazioni analitiche: pertanto utile accettarlo come raccomandazione, convinto che quei principi siano importanti e debbano guidare l'azione del legislatore delegato.

i punti che tratta l'emendamento sono altri e diversi, e pregherei di prenderli in considerazione tutti. Siamo di fronte a una delega per il recepimento della direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. Una direttiva pesante, devo dire, rispetto ai datori di lavoro che consapevolmente assumono e fanno lavorare persone senza permesso di soggiorno, e quindi in condizioni, poi, di lavoro nero:

Noi riteniamo che forse una delega non guidata da alcuni indirizzi possa essere troppo ampia.

infatti del tutto evidente che non possiamo avere una legislazione molto rigorosa per i lavoratori

e credo che uno sforzo comune per individuare alcuni paletti - ne ho indicati, esemplificando, alcuni - sia utile per non fare della comunitaria una specie di grande legge delega in bianco:

che il Governo debba avere la più ampia delega possibile per cercare di recepire la direttiva, coordinandola con le norme già vigenti. Ricordo comunque che si tratta di una delega

il diritto comunitario prevale sempre sul diritto nazionale, che le misure nazionali che lei ritiene così importanti e stringenti, qualora la direttiva entrasse in vigore nel nostro Paese

con questa scelta sbagliata da parte della 5a Commissione si determina un effetto *boomerang* rispetto all'infrazione, cioè un aggravio di spesa per lo Stato, quello sì, per certi versi,

le direttive, è impossibile calcolarne l'esito. Questo problema ha ricadute dal punto di vista economico, ma nel caso della direttiva sul rientro volontario colpisce anche esseri umani.

le armi da guerra esportabili fanno parte delle scelte di politica estera dello Stato italiano. Non si fa riferimento al Parlamento, al Governo e alle singole istituzioni, ma, ripeto, allo Stato italiano. Di conseguenza, vi è un regime di autorizzazione che fa eccezione rispetto alle scelte di mercato individuali delle aziende. Questa legge, che, lo ribadisco, è una delle più avanzate, potrebbe essere presa come riferimento per l'Unione europea.

Saggiamente il sottosegretario Scotti e la Presidenza della Commissione hanno riportato il discorso nei termini delle norme e dei principi sanciti dalla legge n. 185. Credo che il Partito Democratico abbia dato un contributo importante, con gli interventi dei colleghi Scanu e Del

nella legge, e noi riteniamo di riaffermarlo in questa sede perché sia chiaro all'interpretazione successiva. In ogni caso, il Governo conferma l'emendamento 16.500

perché si tratta di una direttiva che ha a che fare con modalità e condizioni dei trasferimenti all'interno dell'Unione europea dei prodotti per la difesa. Una tematica, non solo politicamente, perché ha a che fare con la politica europea di difesa, ma anche perché tratta del delicato tema della circolazione dei materiali di difesa a livello europeo.

la proposta di direttiva nella cosiddetta legge comunitaria di questo anno, sia per i contenuti politici che il testo originale della proposta del Governo aveva.

la legge comunitaria annuale - che la legge n. 11 del 4 febbraio 2005 individua quale strumento normativo cardine, diretto ad assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. L'approvazione della legge comunitaria rappresenta quindi un momento di viva e consapevole partecipazione del Parlamento al processo di integrazione europea, anche per assolvere agli impegni

ma un provvedimento che costituisca uno dei passaggi di maggiore importanza per la nostra partecipazione al processo di integrazione europea: un momento che dovrebbe essere di ampia condivisione e di sintesi tra le diverse componenti

Io ho concluso il mio intervento in discussione generale con un approccio molto positivo per quanto riguardava il voto finale della legge comunitaria. Tuttavia, dobbiamo dire che vi sono stati dei momenti in cui abbiamo registrato una chiusura da parte del Governo su

un emendamento che tutelava un organismo che è fondamentale per garantire pluralismo ed equità nell'informazione.

Era logico attendersi un comportamento più collaborativo da parte del Governo e della maggioranza. Era l'occasione per una più stretta collaborazione, proprio perché si trattava della legge comunitaria, tra maggioranza e opposizione: così, purtroppo, non è stato. Uno dei motivi più rilevanti per cui si è costituito il Gruppo Futuro e Libertà

e di arrivare, attraverso un dibattito libero, alle sintesi di questo e a decisioni condivise. Dico ciò, perché è evidente che, anche in questa occasione,

di verificare l'accoglimento o meno da parte del Governo della nostra risoluzione. un emendamento, riferito alla proposta di risoluzione n. 2 accettata dal Governo, avente come primo firmatario il presidente Viespoli, firmato da tutto il Gruppo di Futuro e Libertà.

Le ragioni le ho illustrate nella discussione generale, le hanno ribadite i colleghi Lannutti e De Toni, in merito ai settori delle telecomunicazioni e del credito finanziario, e le ha confermate la bocciatura delle nostre proposte emendative. Sarò pertanto molto veloce. Ho già detto come il ritardo cronico ormai accumulato non sia più accettabile in un sistema modellato dal Trattato di Lisbona dove si prevedono celerità e flessibilità nell'adeguare il diritto interno a quello comunitario. Questo fatto è la spia, ancora una volta, di quanto il Governo non abbia compreso l'importanza di essere un membro dell'Unione europea, l'importanza delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, la rilevanza degli obblighi che come che come Stato abbiamo nei confronti di Bruxelles. Ci troviamo oggi ad avere i bilanci pubblici praticamente decisi con la nuova *governance* in sede europea, ma ancora non riusciamo a rispettare i tempi dettati per la legge comunitaria dalla legge Buttiglione. Sarebbe già questo un motivo sufficiente per astenersi. come il Governo dimentichi, di anno in anno, le posizioni emerse durante la discussione della precedente legge comunitaria. tutte quelle osservazioni fatte, da maggioranza e opposizione, nei confronti della legge comunitaria 2009, sono state azzerate e disattese in questa proposta normativa per il 2010, nonostante ci fossero stati degli impegni da parte del Governo ad ascoltare le riflessioni parlamentari nella successiva sessione comunitaria. Questo oblio è calato sia sugli aspetti tecnici che su quelli politici, dei quali un esempio su tutti è la direttiva che sanziona i datori di lavoro degli immigrati illegali. Una dura battaglia aveva portato le opposizioni a votare contro la legge comunitaria un anno fa proprio perché la stessa non recepiva la direttiva in questione. Ci aspettavamo che almeno questa volta, nella seconda possibilità offertaci, venissero rispettate e accolte le richieste avanzate da chi vuole tutelare l'immigrazione legale e punire chi si arricchisce con quella illegale, ma purtroppo niente di tutto questo. Gli immigrati rimarranno stretti fra decreti flussi insufficienti ed il caporalato. Per questo continuo spregio dell'opposizione, su una legge come la comunitaria che dovrebbe vedere invece il consenso *bipartisan*, l'Italia dei Valori si asterrà. La legge contiene inoltre disposizioni su cui non possiamo essere d'accordo, poiché sono state inserite in maniera autoritativa nella legge comunitaria quando avrebbero dovuto essere oggetto di una riflessione a parte con un provvedimento autonomo e analizzato dalle Commissioni competenti. Innanzitutto la disposizione sulle armi, la cui illegittimità, per il metodo usato in principio, ci ha fortemente indignato, riuscendo solo dopo lunghe trattative ad ottenere un parziale ripristino del rispetto del ruolo del Parlamento. Ma anche la disposizione su Roma capitale, che crea uno *status* della capitale senza nessuna determinazione dei poteri e delle funzioni, è una forzatura che ignora quanto sta facendo la Commissione bicamerale per il federalismo fiscale. Ma ci vede anche contrari la disposizione sull'istituto della fiducia all'articolo 11. Infine non posso non sottolineare come un Governo senza Ministro per le politiche sia un Governo che non ha titoli per portare avanti l'importante percorso dell'integrazione comunitaria, e nemmeno per licenziare e vedersi approvate da noi, leggi comunitarie senza alcun padre nobile. Sul sito del Governo alla voce Ministri e Ministeri, accanto alla voce «Ministro per le politiche europee», ci sono tre desolanti punti di sospensione, che dal 15 novembre rappresentano per gli osservatori internazionali la nostra vergogna. Questo è il valore che il nostro Esecutivo dà all'Unione europea: si approverà una legge comunitaria senza che vi sia un esponente del Governo responsabile per il provvedimento. È assolutamente inconcepibile, colleghi. con molta disponibilità, estrema competenza e profonda attenzione ha seguito tutta l'analisi del disegno di legge in Commissione, ma è un Sottosegretario "prestato" dal Ministero degli affari esteri, se il presidente Berlusconi, ed è lui che, gioco forza, avrebbe dovuto impegnarsi in prima persona, poiché è l'unico formalmente responsabile per il Governo rispetto alla legge comunitaria. Tuttavia il "Presidente del Consiglio che non c'è" non si è mai presentato in Commissione e manca anche oggi in Aula. Nella proposta di risoluzione presentata dall'Italia dei Valori in merito alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia alla Unione europea abbiamo chiesto che il Governo si impegni a nominare, nel più breve tempo possibile, il nuovo titolare del Ministero per le politiche europee, al fine di garantire operatività al Dipartimento per le politiche comunitarie e piena rappresentanza al nostro Paese in seno alle istituzioni europee in quanto la vacanza di tale carica ha comportato l'affidamento *ad* *interim* ad una persona (ripeto), il Presidente del Consiglio, che in questi mesi non ha mosso un passo per l'Unione europea, avendo già rilevanti impegni per la carica che ricopre, oltre agli impegni legati alla sua personalissima battaglia per sottrarsi alla giustizia nella bufera giudiziaria e negli scandali che lo hanno investito. Abbiamo anche chiesto che venga garantito il rispetto dei tempi previsti per la presentazione al Parlamento della relazione annuale per il 2010 e della legge comunitaria per il 2011; che si giunga ad una efficiente ed efficace *governance* economica, riformando in tempi brevi la procedura di bilancio alle linee guida sancite a livello europeo; che vengano potenziati i risultati ottenuti sia in merito alla riduzione del numero di procedure di infrazione, allineando il dato attuale (123 procedure aperte) con quello inferiore degli altri Paesi dell'Unione europea, sia del *deficit* di trasposizione delle direttive comunitarie, passando da un *deficit* dell'1,4 per cento all'1 abbiamo chiesto inoltre che vengano rafforzati i poteri della 14a Commissione, al fine di trasformarla da Commissione subordinata alle altre in organismo proponente per l'elaborazione delle normative comunitarie e giudicante in ultima istanza nella trasposizione delle delle stesse nel nostro ordinamento. Sappiamo già che tutto ciò sarà disatteso, così come non ci aspettiamo niente di positivo sul piano delle nomine, che risponderanno come ogni volta a calcoli di alleanze o a interessi personali del Premier (come ha insegnato il caso Romani al Ministero dello sviluppo Lo sappiamo perché già durante l'analisi della legge comunitaria 2009 abbiamo chiuso con auspici che sono stati puntualmente, purtroppo, dimenticati. Cari colleghi, signor Presidente, come Assemblea legislativa abbiamo perso la nostra capacità di indirizzo programmatico nei confronti del Governo rispetto alla politica e alle posizioni da tenere nelle sedi dell'Unione europea. Il Parlamento nazionale partecipa tanto e bene nella fase ascendente, ma lo fa solo con riguardo al rapporto diretto che ha instaurato con la Commissione europea, mentre i suggerimenti e le obiezioni con l'interlocutore più naturale, il Governo, vengono vanificati perché non ci sono spazi formali per farlo: la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è ancora più vecchia della legge comunitaria, e la nuova relazione, quella programmatica che il Governo dovrebbe presentare a seguito delle modifiche alla legge Buttiglione, giace sulla scrivania del Ministero perché manca il Ministro competente. Questo dialogo Parlamento-Commissione e il silenzio Parlamento-Governo è un assurdo è un assurdo istituzionale. Come Italia dei Valori, in conclusione, chiediamo una inversione di rotta e sulla legge comunitaria così

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, siamo oggi chiamati a licenziare la legge comunitaria 2010 arrivata in Parlamento all'inizio dell'agosto 2010. Come sempre, siamo in forte ritardo sulla tabella di marcia. Basti pensare che entro lunedì scorso, il 31 gennaio, si sarebbe dovuta presentare la comunitaria per il 2011. L'assenza del Ministro di riferimento, dal 15 novembre scorso, giorno in cui il ministro Ronchi ha rassegnato le sue dimissioni, ha sicuramente aggravato ulteriormente il grosso problema della tempistica. Il vero problema, oltre alla tempistica del Parlamento, è l'inadempienza delle amministrazioni a cui spetta confezionare i decreti attuativi delle direttive. Il secondo problema che ne deriva riguarda le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia e tuttora pendenti. Voglio ricordare che solo la settimana scorsa l'Unione europea ha aperto altre 24 nuove procedure di infrazione, di cui una buona parte riguarda direttive contenute nella legge comunitaria 2009 e per le quali i decreti di attuazione sono ancora mancanti. Queste 24 nuove procedure di infrazione si aggiungono alle 24 preesistenti tutte per mancata attuazione delle direttive nell'ordinamento italiano. Inoltre pesano le 96 procedure di infrazione aperte per violazione del diritto comunitario; pertanto risultano ad oggi aperte, nei confronti del nostro Paese, 144 procedure di infrazione per la mancata o non corretta attuazione delle direttive comunitarie. Dobbiamo assolutamente accorciare i tempi; si potrebbe ad esempio, come fanno gli altri Paesi europei, iniziare l'*iter* di recepimento durante le fasi di conclusione della direttiva. I settori che sono oggetto del maggior numero di infrazioni sono quelli dell'ambiente, della salute, dei trasporti e della fiscalità e dogane, del lavoro e degli affari sociali. Cresce anche il numero delle lettere di messa in mora e quello delle sentenze di condanna emesse in primo grado dalla Corte di giustizia europea. Le prime salgono infatti da 73 di due anni fa a 79, mentre le decisioni sfavorevoli della Corte sono passate da 10 a 12. La definitività delle condanne esporrebbe il nostro Paese a pesanti sanzioni pecuniarie. Dobbiamo essere concordi una volta per tutte sul fatto che l'Italia non può permettersi condanne onerose per la finanza pubblica. Queste risorse ci servono per ben per altre cose! Prima di entrare nel merito del provvedimento vorrei ringraziare la presidente della 14a Commissione e relatrice di questo provvedimento, senatrice Rossana Boldi, per il proficuo lavoro svolto in Commissione. Innanzitutto, tengo a mettere in risalto l'articolo 5 che conferisce una delega al Governo per l'emanazione di testi unici e codici di settore riguardanti le disposizioni comunitarie, dettate in attuazione delle direttive stesse al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative, vigenti nelle stesse materie. La delega rappresenta un ottimo strumento per operare periodicamente un coordinamento e riordino del sistema normativo. Significativo è altresì l'articolo 6 sulla registrazione dei dispositivi medici con il quale si elimina l'obbligo di pagamento di 100 euro per ogni registrazione effettuata nel repertorio dei dispositivi stessi. L'articolo 8 recepisce le novità europee sul fronte degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari rispetto a quelli di origine. Le modifiche normative proposte sono necessarie per avviare in Italia il pieno funzionamento del cosiddetto passaporto delle società di gestione del risparmio che ora permette a queste ultime di costituire fondi comuni in un Paese membro dell'Unione europea diverso da quello di origine. Oltre a ridefinire l'operatività transfrontaliera, vengono attribuite a CONSOB e Banca d'Italia i poteri di vigilanza e d'indagine che la direttiva prevede. Compie un passo in avanti il riordino della professione di guida turistica. L'articolo 10, infatti, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino di tale professione, disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio. In particolare, con il decreto dovranno essere individuati dei requisiti minimi per l'accesso alla professione e un percorso formativo oltre che indicati i requisiti generali da approfondire poi in sede di disciplina regionale, al fine di adeguarli alle peculiarità territoriali. Attualmente, esiste un irragionevole regime di discriminazione nei confronti dei cittadini italiani, dato che l'esercizio dell'attività delle guide italiane continua ad essere vincolato al territorio regionale o provinciale in cui sono abilitate, mentre le guide straniere che intendono intendono svolgere un'attività anche sul nostro territorio nazionale sono tenute unicamente ad una informativa preventiva. Con un importante modifica apportata dalla 14a Commissione, in sede referente, si è introdotto il requisito per cui l'esercizio della delega avverrà nel rispetto degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Nell'articolo 11 troviamo il cosiddetto pacchetto Telecom con cui vengono recepite le direttive dell'Unione europea che mirano a rafforzare i diritti degli utenti telefonici e di Internet e ad incoraggiare la concorrenza fra gli operatori del settore delle telecomunicazioni. Ho elencato fin qui le misure della legge comunitaria 2010 che ritengo più significative. Adesso il provvedimento passerà all'esame dell'altro ramo del Parlamento e auspico che mantenga i contenuti propri della legge comunitaria anziché trasformarsi in maniera impropria e strumentale, in un contenitore di disposizioni eterogenee.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il disegno di legge che stiamo per approvare reca le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. La legge comunitaria è il principale strumento di adeguamento dell'ordinamento interno agli indirizzi europei che, come ogni anno, conferisce al Governo le deleghe necessarie a recepire nell'ordinamento nazionale le direttive emanate dall'Unione europea con criteri generali e specifici per talune materie. Questa legge comunitaria, grazie alla collaborazione di tutti i membri della 14a Commissione che si sono attenuti in modo scrupoloso ai rigorosi criteri di ammissibilità degli emendamenti fissati, si presenta con un testo "snello", privo di disposizioni che non attengono all'oggetto tipico della legge stessa. Abbiamo, tutti insieme, evitato che le proposte emendative trasformassero il disegno di legge in un improprio provvedimento *omnibus*. Indubbiamente pesa la mancanza di un Ministro di riferimento. Non solo. A mio avviso diventa sempre più indispensabile una riforma del Regolamento del Senato che preveda un esame disgiunto del disegno di legge comunitaria rispetto alla Relazione annuale sulla partecipazione all'Unione europea. E ancora, sarebbe opportuno ampliare i casi di esame in sede referente per la 14a Commissione anche a quei provvedimenti che presentano un contenuto analogo a quello della legge comunitaria o che abbiano un contenuto eterogeneo e siano finalizzati alla necessaria attuazione di obblighi comunitari, come per esempio quelli previsti dall'articolo 10 della legge n. 11, del 2005 i cosiddetti provvedimenti salva-infrazioni. La necessità di adeguare l'ordinamento interno alle innovazioni apportate dal Trattato di Lisbona, richiede una riforma dello strumento della legge comunitaria, passaggio che giustifica la presenza di diverse proposte di modifica della legge Buttiglione e del disegno di legge governativo ora all'esame della XIV Commissione della Camera dei deputati. Non voglio entrare nel merito delle diverse proposte di modifica della legge Buttiglione, non è questa la sede, certamente esse mirano alla predisposizione in tempi brevi

La Lega Nord esprime apprezzamento per il contenuto della legge che andiamo ad approvare e si augura che nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento, essa non si ritrasformi di nuovo in un contenitore per ulteriori e disomogenee disposizioni. Riferendomi al contenuto della legge che oggi andiamo ad approvare, vorrei porre in evidenza alcuni passaggi che la Lega Nord ritiene di dover segnalare. Primo fra tutti, ed è già previsto dall'articolato, la precisazione che in relazione ai testi unici o ai codici di settore riguardanti principi fondamentali nelle materie di cui

La Lega Nord ritiene che ciò debba essere consolidato e valorizzato anche attraverso la partecipazione più incisiva delle Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea fin dalla fase ascendente. Il secondo è quello relativo all'articolo 10 che riguarda il riordino della professione di guida turistica che non andrà a compromettere i percorsi formativi relativi alla conoscenza di specifiche aree del territorio nazionale particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale e ambientale. Ben venga il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo delle Regioni e delle Province autonome quali soggetti istituzionali per definire i percorsi formativi per le guide turistiche. Per concludere, la Lega Nord e convinta della qualità del lavoro svolto su questa legge comunitaria e per questo è doveroso ringraziare la presidente della Commissione, nonché relatrice, senatrice Boldi, i colleghi della Commissione ed il Governo, che ha garantito la sua presenza nei passaggi fondamentali della fase emendativa sia in Commissione che in Aula. Si tratta di un provvedimento di rilievo ed innovativo, come già spiegato, certamente importante per un'attiva partecipazione dell'Italia al processo di integrazione comunitaria ed è per questo che il Gruppo della Lega Nord voterà a favore di questo

della vergognosa legge approvata l'anno passato (una legge nata con 11 articoli e finita con 55 articoli, all'interno dei quali erano state inserite norme che potevano stare tranquillamente nel cosiddetto milleproroghe o in altri provvedimenti), almeno questa legge, come noi abbiamo chiesto più volte in questa legislatura, si limita a materie che riguardano la legge comunitaria, con qualche piccolo scivolone (è stato già detto) come il tentativo di cambiare la legge sul commercio delle armi, una delle più avanzate in Europa, tramite un emendamento di cinque pagine (alla fine saggiamente ritirato dal Governo grazie alle pressioni del Partito Democratico) qui dentro (per esempio quella della professione forense, che è andata contro la richiesta dell'Unione europea), poteva anche essere inserita in un altro provvedimento. Tuttavia, se è vero che la legge comunitaria certamente è una moneta a due facce, però guardare anche la faccia della normalità del successo. La normalità dell'Europa, che possiamo criticare, è anche indice del successo dell'idea dell'Europa: di un'Europa in cui 27 Paesi vivono senza conflitti (alcuni da più di 65 anni) ed a cui altri hanno aderito proprio perché hanno subito un conflitto negli anni

per l'Europa federale e solidale. L'Europa è la normalità. L'Europa la si può criticare, ma lo si può fare perché esiste. E in questa Europa il problema è rappresentato dal ruolo dell'Italia. Vorrei dire sommessamente - perché è presente in quest'Aula, e la stimo molto che un Ministro di un Governo precedente aveva ridotto il livello di non recepimento delle direttive all'1,4 superando di molto anche la percentuale raggiunta in questi tre anni, in cui pure noi abbiamo collaborato

la possibilità di rimpatrio volontario, in cui si enfatizza, nelle sole tre righe che sono state approvate, l'allungamento dei tempi del CIE in Italia

per motivi di campagna elettorale e andando contro il federalismo e contro le scelte che dovrebbe fare un Governo in tema di sicurezza (quindi, contro la sicurezza dei cittadini),

divenga un meccanismo di stabilità serio, con un Ministro del tesoro. Abbiamo fatto la scelta europea di avere un servizio diplomatico europeo,

del tesoro a livello europeo. Abbiamo già la Banca; non bastano gli *eurobond* (su questo Tremonti ha ragione), dobbiamo avere un governo della stabilità economica, e questo significa riformare il Patto di stabilità e migliorare la concertazione.

È evidente che l'Europa ha bisogno di fatti, non possiamo dividerci per questioni italiane. Dobbiamo semmai dividerci e confrontarci, come è giusto, su questioni europee. Sono i fatti che ci dicono se siamo europei o no.

voi, dovremmo cercare quelle che lo scrittore Amin Maalouf ha definito le origini? Le radici sono nel terreno, sono segrete, tengono l'albero prigioniero; le origini appartengono a tutti noi, riguardano i ragionamenti sulla vita e la morte di Ingmar Bergman o il provvidenzialismo di Manzoni, ma anche il Bertoldo, che

In primo luogo, però, desidero sinceramente ringraziare la senatrice Boldi e il senatore De Eccher per avere curato questi documenti finalmente nella forma che tutti andavamo auspicando da anni, vale a dire in forma semplificata e soprattutto facile anche da discutere. È stato detto più volte, quindi in sede

Va detto che non siamo ancora arrivati al punto che vorremmo, in quanto dovremmo riuscire a dibattere questa legge entro il 31 dicembre dell'anno di esercizio: siamo nel mese di febbraio, per cui avremmo dovuto già avere in mano la comunitaria del 2011. Ci stiamo però arrivando, un po' alla volta. Questa volta. Questa aspirazione non è un puro esercizio di rapidità operativa o di semplificazione, ma risponde all'esigenza primaria di scongiurare per l'Italia nuove procedure di infrazione comunitaria: infatti, la ritardata applicazione di una direttiva produce questi effetti.

un paio d'anni siamo scesi dal primo al sesto posto della graduatoria: ciò significa che è in atto un percorso virtuoso di recupero, e molto dipenderà anche dalle prossime comunitarie. Sui vari senatori si sono soffermati, e sarebbe lungo farlo anche in questa sede. Desidero però segnalare la felice soluzione dell'articolo 16, che parla di prodotti d'arma,

alla popolazione, quali le acque di balneazione, le comunicazioni elettroniche e la professione di guida turistica. Vorrei segnalare, nel campo del lavoro e della previdenza, l'articolo che prevede una informazione dei lavoratori sulle aziende transnazionali e poi ancora quello che si occupa di prodotti magistrali, anticamera di un disegno presente al Consiglio d'Europa, che vorrebbe introdurre il reato di crimine farmaceutico. Per l'istruzione e la cultura, fra le molte iniziative

Per il settore agricolo non vi sono grandi innovazioni, salvo il fatto di occuparci di biotecnologie e organismi geneticamente modificati. Sono adempimenti che dovrebbero porre l'Italia alla pari degli altri Paesi europei, per cui non si tratta di anticipare i tempi, ma di recuperare una posizione che ancora non è ottimale. dire anche in questa sede - sono d'accordo con coloro che lo hanno ricordato, penso in particolare alla collega Bonino - che saremmo in colpa se ci lasciassimo sfuggire l'opportunità di allargare il dialogo sullo stato di salute dell'Italia in Europa e dell'Unione europea nel suo insieme. La legge comunitaria dovrebbe proprio essere riscattata da questo ruolo di occasione formale, formale, burocratica, per contenere spunti di riflessione più generale. Vi è un aspetto molto importante per il futuro. Il nuovo Trattato di Lisbona attribuisce alle Commissioni per le politiche comunitarie nuove prerogative in fase ascendente, soprattutto per la correzione delle proposte di direttive e di normative che provengono dalla Commissione europea. europea. La nostra Commissione si è particolarmente impegnata: in una graduatoria reale che esiste fra i Parlamenti europei è ai primissimi posti. Questo non significa la ricerca di una *leadership* banale,

ma anche nel merito delle iniziative legislative. Faccio una proposta, che è molto simile ad una provocazione, e me ne assumo la paternità: questo dovrebbe portare ad una rivisitazione anche dei rapporti tra la 14a Commissione e le altre Commissioni permanenti del Senato.

parere. È un'inversione dei ruoli importante, perché darebbe alla Commissione per le politiche europee nuova dignità, ma soprattutto rispetto del Trattato di Lisbona e delle nuove attribuzioni. Faccio, infine, un accenno all'Europa politica e ai La cosiddetta legge comunitaria, lo abbiamo detto, dovrebbe essere l'occasione anche per cercare di capire dove stiamo andando noi, come italiani, in Europa, ma soprattutto dove stia andando il sodalizio europeo, nel concerto delle altre grandi organizzazioni mondiali. Molte contraddizioni sono evidenti e sono all'ordine del giorno, questo era previsto fin dall'origine; non a caso Robert Schumann, uno dei padri dell'attuale Unione europea, diceva: «L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto». Possiamo dire che dopo 54 anni questa solidarietà di fatto ancora non vi sia, e dal Trattato di Roma ad oggi molti altri trattati hanno riformato gli spiriti comunitari. La dimostrazione è venuta proprio l'altro ieri nell'episodio che ha ricordato il collega Di Giovan Paolo, quando,

per segnalare una recrudescenza nel mondo molto pericolosa ed evidente di persecuzioni mirate verso le comunità cristiane. Ne abbiamo parlato anche al Consiglio d'Europa citando dettagliatamente caso per caso. Nell'ultimo anno, nel mondo sono stati uccisi 2.166 cristiani, in una serie sterminata di incursioni e razzie. Abbiamo saputo che questa iniziativa non solo italiana, non ha trovato il necessario appoggio: era stata suggerita per l'approvazione una formulazione ipocrita, che voleva sostituire la definizione di comunità cristiana con comunità religiosa. È un tentativo non nuovo in Europa: basti ricordare la lotta per il preambolo della Costituzione che, invece, di contemplare le radici cristiane menziona radici religiose.

Al Consiglio d'Europa, invece, un analogo documento è stato approvato da 47 Paesi, molti dei quali di radici musulmane e islamiche. il documento, tranne la Turchia, che si è astenuta perché un emendamento non è stato eliminato. Questo ci dovrebbe far riflettere su dove stiamo andando in Europa con il sodalizio dell'Unione europea: perché in un'Assemblea di 47 Paesi, con Paesi caucasici e balcanici, si riesce a trovare la coesione su un tema così delicato e importante, e non si trova tra i 27 Paesi dell'Unione europea? Tento una risposta, signor Ministro: è a causa dell'elevato tasso politico del Consiglio europeo, a differenza del Consiglio d'Europa che ha differenti obiettivi? mettendo le manette ai Ministri degli esteri o di altri Dicasteri, rallenta il processo di coesione? Va detto però che il ministro Frattini, che si è battuto fino all'ultimo, ha già annunciato che ripresenterà un documento simile in una prossima occasione. È quindi quindi con amarezza che dobbiamo ancora una volta constatare che la cosiddetta politica estera europea è un'utopia e che il cosiddetto Alto rappresentante della politica estera europea, la signora Ashton, Ashton, si rivela ad ogni prova delicata sempre più inadeguata al ruolo in cui è stata collocata. Anche qui, però, nulla di nuovo, e direi anche nulla di preoccupante. Del resto, lo diceva Jean Monnet, un altro dei grandi padri dell'Unione europea:

è presente in tribuna una delegazione di studenti del Liceo scientifico «Carlo Levi» di Irsina, in provincia di Matera. A loro va il saluto dell'Assemblea. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo

in particolare, al contenuto di proposte di legge già depositate presso il Senato della Repubblica, proposte che evidentemente non si conoscono nel dettaglio e che potrebbero essere teoricamente tra di loro, non solo distanti, ma addirittura incompatibili o contraddittorie.

tuttavia mi sarei atteso semmai una richiesta di riformulazione, perché è evidente che l'obiettivo politico dell'emendamento è quello di sottolineare l'esigenza di affrontare - come dovrebbe essere negli auspici di qualsiasi Governo

del senatore Menardi, che va esattamente nella direzione del recepimento della direttiva e dell'esigenza di un raccordo. In effetti, il primo modo per dare una frustata, non al cavallo, ma all'intelligenza creativa ed imprenditoriale di questo Paese, è quello di determinare le condizioni perché le pubbliche amministrazioni paghino in tempi ragionevoli. Non riesco a capire perché mai questo ovvio questo ovvio obiettivo di buonsenso e di qualità di governo trovi una sorta di burocratico - per non dire altro! - impedimento, che è solo pregiudiziale, e che riguarda quindi il pregiudizio e non il giudizio. Presidente Viespoli, mi è sembrato di capire, dall'intervento del senatore De Eccher, che il nodo sta nel riferimento ai provvedimenti legislativi.

Presidente, vorrei pregare il senatore Viespoli di cogliere l'indicazione che il relatore ha offerto, cioè convergere sulla sostanza della proposta in termini di un ordine del giorno, che il Governo accoglierebbe. Presidente, io comprendo il senso della riflessione e dell'invito del sottosegretario Scotti. però, signor Sottosegretario, il motivo per il quale non si possa integrare la risoluzione con un riferimento al recepimento di una direttiva europea, determinando così la condizione per fare riferimento alle iniziative che il Parlamento riterrà di assumere, compatibilmente con la linea e con l'impostazione. In caso contrario, non vi è alcun problema. Voteremo l'emendamento e prenderemo atto della qualità del confronto e del dibattito parlamentare.

Colleghi, avete votato tutti?

Con l'approvazione del disegno di legge n. 2322 e della proposta di risoluzione n. 2 si intende esaurita la discussione della Relazione all'ordine del giorno.

La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca: «Votazione sulle dimissioni presentate dai senatori Salvatore Cuffaro e Nicola Rossi». Con lettera pervenuta alla Presidenza in data 31 gennaio 2011, il senatore Cuffaro ha comunicato di rassegnare le proprie dimissioni da senatore della Repubblica.

Libertà voterà contro le dimissioni del collega Nicola Rossi. Lo farà per tenere fede ad una consuetudine che in quest'Aula c'è sempre stata:

imparato ad apprezzare l'indipendenza di spirito e la capacità critica, pur espresse con un comportamento che è sempre stato disciplinato

Credo che le buone tradizioni in quest'Aula non debbano essere abbandonate, e tra le buone tradizioni c'è anche quella per la quale, se non per gravi motivi, una prima una prima votazione deve essere un segno di stima che si manifesta con un voto contrario. differenti, quelle ragioni eccezionali alle quali ho fatto riferimento, ci porteranno invece a votare a favore, come Gruppo del PdL, delle dimissioni del collega Salvatore Cuffaro. Se non ci fossero queste dimissioni, per la vicenda giudiziaria che ha visto Cuffaro protagonista, ci sarebbe la decadenza

molto sobria. Una prima è una ragione personale, che però interpreta i sentimenti di una parte ampia di questo Gruppo: per l'amicizia che molti di noi hanno nei confronti di Salvatore Cuffaro, che si testimonia anche e soprattutto nei momenti di sorte avversa.

concorso esterno al favoreggiamento aggravato, dal punto di vista garantistico non ha migliorato la situazione, soprattutto se si tiene conto dello iato che passa tra le richieste del procuratore generale e la sentenza. Il terzo motivo è prettamente umano. È la stima per come Cuffaro si è comportato in questa vicenda, per come ha accettato la sua sentenza. Tutto ciò non merita una decadenza, ma che l'esito della sua vicenda parlamentare sia deciso da lui attraverso le dimissioni liberamente offerte. *(Applausi dal

che condividiamo in gran parte, nella sostanza. La decisione del Gruppo è in relazione all'opportunità che si eviti la decadenza e si accompagni la scelta che il senatore Cuffaro ha ritenuto di fare.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi voteremo a favore delle dimissioni del senatore Cuffaro, e riteniamo che, in fondo, le sue dimissioni abbiano evitato a quest'Aula di pronunziarsi utilizzando un istituto indubbiamente sgradevole qual è quello della decadenza. In questo, condivido la riflessione del senatore Quagliariello. la Camera alta o qualunque altra istituzione, ma specie la Camera alta, è costretta a pronunziarsi sulla decadenza di un proprio componente, è una pagina triste. Indubbiamente, le dimissioni hanno evitato a quest'Aula di doversi pronunziare attraverso questa formula così draconiana. Non mi aspettavo, a dire la verità, che si cogliesse quest'occasione, in cui responsabilmente noi prendiamo atto del fatto che si sia evitato di scrivere una pagina triste per il Senato, per definire la giurisprudenza di 29 anni in materia di

anche la pedopornografia, anche la prostituzione minorile. In realtà, esistono categorie del diritto codificate ed interpretate dalla giurisprudenza.

Rammento che il reato è previsto dal nostro codice e che su quel reato, previsto dal nostro codice, attraverso una combinazione di più articoli, si è solidificata, sedimentata e sviluppata una giurisprudenza di oltre 29 anni. Signor Presidente, noi voteremo per l'accoglimento delle dimissioni del collega Cuffaro

rispetto al fatto che l'Aula si pronunci preventivamente sull'istanza che viene dal collega senatore che intende lasciare l'incarico. Il secondo è che intendiamo rispettare la decisione che il senatore Cuffaro ha inteso porre in essere, come atto consequenziale di rispetto

dare corso all'esecuzione del provvedimento giudiziario, ivi comprese le dimissioni da componente del Senato. Credo sia un comportamento che molti dovrebbero imitare, perché c'è bisogno di serenità e rispetto delle istituzioni, anche quando queste possono adottare scelte criticabili,

ci hanno visto divisi rispetto ai progetti futuri. Questa è la ragione per la quale, anche per affetto e rispetto personale, ma soprattutto per rispetto della scelta che ha fatto, noi accoglieremo le sue dimissioni.

con il senatore Cuffaro hanno un rapporto affettivo importante. Per questa ragione voglio rispettarne integralmente le indicazioni, avendo preso atto di un sentimento diffuso, anche di apprezzamento, che ha superato gli schieramenti, rispetto ad un comportamento

davvero opportuna la notazione del collega Viespoli secondo cui è molto più rispondente, se si vuole attestare stima e apprezzamento per questo comportamento rigoroso del senatore Cuffaro, procedere con l'accoglimento delle dimissioni piuttosto che perfezionare un istituto sgradevole qual è quello della decadenza. In questo senso, anche i senatori del mio Gruppo voteranno per l'accoglimento delle dimissioni del senatore Cuffaro.

porre una questione. Nel nostro codice di procedura penale c'è scritto che un cittadino può essere condannato soltanto se il giudice lo ritiene colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. In primo grado, in nome del popolo italiano, il nostro collega Cuffaro era stato riconosciuto innocente e prosciolto in ordine all'aggravante di aver favorito la mafia. Viceversa, in appello (cartaceo, senza un dibattito) è stata poi riconosciuta la sua colpevolezza. quindi arrivati in Cassazione, e il procuratore generale della Cassazione, cioè l'accusa, ha affermato che non esisteva alcuna prova che il senatore Cuffaro avesse mai favorito la mafia:

e all'università mi insegnavano che *in dubio pro reo*. Nella norma c'è scritto: «al di là di ogni ragionevole dubbio»: ma io sono pieno di dubbi. in questo caso siamo al di qua e non al di là di ogni ragionevole dubbio, ed è un problema, questo, che riguarda tutti i cittadini italiani e il nostro sistema processuale, tant'è vero che nella precedente legislatura - lo dico ad alcuni colleghi - era stata già fatta una riforma che prevedeva che non si mettesse in contraddizione il popolo italiano con se stesso, specialmente quando una persona viene prosciolta e si gioca la vita in una specie di partita di tennis, che può finire 1 a 2

(e la penso come il tribunale di primo grado e come il procuratore generale della Cassazione), se permettete, credo che il Senato e la Camera, rispetto a ogni cittadino italiano, dovrebbero porsi il problema di cosa voglia dire quando un cittadino sta anni e anni in galera, al di là di ogni ragionevole dubbio, quando gli stessi giudici e gli stessi magistrati hanno espresso con le assoluzioni su quel punto i loro dubbi sulla sua colpevolezza, come nel caso del senatore Cuffaro.

I senatori favorevoli ad accogliere le dimissioni premeranno il tasto verde al centro della postazione di voto; i senatori contrari premeranno il tasto rosso a destra; i senatori che intendono astenersi premeranno il tasto bianco a sinistra. Poiché si tratta di una votazione a scrutinio segreto, qualunque sia la scelta di voto effettuata, la luce che si accenderà sarà di colore neutro. Dichiaro aperta la votazione.

Signor Presidente, il nostro voto sarà volto a respingere le richieste del senatore Nicola Rossi, e non per ragioni di cortesia: le nostre sono ragioni di merito ed istituzionali. Noi crediamo che Nicola Rossi, senatore della Repubblica, sia utile alle istituzioni, al suo Gruppo e al Senato, comunque. Riteniamo di compiere un gesto che probabilmente gli dispiacerà, ma che consentirà a lui di rimeditare la decisione che ha assunto, che apprezziamo nella sua linearità (così rara, purtroppo, nei comportamenti pubblici), ma riteniamo che il suo sia un errore e che il suo allontanarsi da questa Aula e rinunciare alla carica di senatore non farebbe né migliore il Senato della Repubblica, né più interessanti e colti i nostri lavori, né più vicino all'esigenza dei cittadini il prodotto del nostro sforzo. *(Applausi

è un onore per me poter dire di essere collega del professor Nicola Rossi. Tanto è vero che quando

Pertanto, riteniamo che le sue dimissioni siano da respingere. Qui si fanno le leggi. Il Senato è la fabbrica delle leggi, la più alta espressione della delega democratica, non esiste fabbrica che rinunci ad uno dei suoi consulenti più esperti. Invito, dunque, il collega Nicola Rossi a ripensarci, a ritirare le dimissioni anche perché le motivazioni non convincono: Nicola Rossi sarebbe qui con qualsiasi legge elettorale.

allora che, proprio per questo motivo, Nicola Rossi debba ritirare le sue dimissioni: per continuare, aapunto a dare un contributo di idee, di intelligenza, di qualità. Lo dico non solo come rappresentante di un Gruppo,

hanno apprezzato questo taglio, questa impostazione, questa capacità. Credo che il Senato non debba privarsi del suo contributo, e perciò voteremo con convinzione contro le dimissioni presentate da Nicola Rossi, anzi con l'auspicio

il nostro Gruppo si pronuncia contro le dimissioni del collega Nicola Rossi, in nome di un principio essenziale, che è quello del contributo del libero intendimento individuale, che i senatori devono dare e che il nostro collega ha già dato ha già dato in passato, anche con ruoli istituzionali di livello. Onestà intellettuale e indipendenza di giudizio sono caratteri che dovrebbero superare il disincanto che immagino il collega abbia verso il suo ruolo attuale, questo senso di limitatezza dovuto alla convinzione di essere nominati invece che eletti. Bisogna dare per superato questo momento, che pure ha una sua potenza; è una questione su cui dovremmo ragionare criticamente sempre, non per prendere la decisione di andarcene, per prendere piuttosto ciascuno la decisione di esercitare le proprie indubbie capacità proprio per cambiare questo quadro che si considera critico. che hanno la vocazione naturale all'indipendenza di giudizio se ne vanno, il rischio è che si inauguri una fase in cui si favorisce piuttosto il predominio del conformismo e della mancanza di iniziativa intellettuale. È perciò con questa idea che il nostro Gruppo respinge le dimissioni Signor Presidente, il Popolo della Libertà conferma il voto contrario alle dimissioni del senatore Nicola Rossi, come già annunciato poc'anzi dal senatore Quagliariello, per la cortesia istituzionale, ricordata appunto dal nostro Capogruppo, per quel garbo istituzionale che ci è molto caro e - aggiungo - anche per qualche motivo sostanziale legato alle sue idee, professor Rossi,

e politica ma anche - l'ha sempre avuta - di anteporre l'interesse generale del futuro del Paese al presente di questo Paese. in nome di quel futuro che noi la invitiamo non a ripensarci, perché non ha bisogno di farlo - Nicola Rossi ha senz'altro meditato, come tutte le sue scelte, anche questa - ma a non

Proprio per evitare la retorica, che so che piace poco al collega Rossi, intervengo solo per testimoniare la stima di un impegno politico e parlamentare fatto di coerenza, di battaglie chiare e lineari, a volte anche poco gradite dalla sua stessa parte politica. Questo la dice tutta sul fatto che ha sempre esercitato con onore ed autonomia il mandato parlamentare, come forse pochi altri hanno fatto in detta legislatura. Questa è la ragione per cui voteremo contro le sue dimissioni.

Mi sento nominato e per questo sento la mia indipendenza limitata. Non ho altra scelta che riprendermi la libertà riconsegnando la nomina».

È vero, perché la legge lo prevede. Non è interamente vero, perché ciascuno dei parlamentari immagina di dare un contributo alla formazione del consenso che poi si deposita nei partiti e nelle liste elettorali. Va anche detto che non è del tutto vero che un meccanismo di collegi uninominali, quale che sia la legge elettorale, non contenga il rovescio di questa medaglia, Presidente, ossia che alla fine ci sia un elemento di scelta per il candidato ma prevalga la scelta per il

per numeri molto piccoli, è bastato che un paio di senatori spostassero la loro posizione, dalla maggioranza alle opposizioni o viceversa, per cambiare la sorte della legislatura.

delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Infatti, un Parlamento fatto di persone che si sentono troppo condizionate dal livello della nomina politica, anziché da quello di una libera dialettica politica che esercitano nei loro partiti, nella coalizione di cui fanno parte e nella relazione con l'opinione pubblica, è un Parlamento che cambia di segno, di natura, di legittimità, di autorità e di autorevolezza. Ecco perché reputo che questa sia forse la prima occasione in cui si discute di motivazioni

crudezza nell'Aula del Senato. Presidente, il punto di fondo è: chi può presentare agli elettori le ragioni di un dissenso politico, misurandole con un consenso

È chiaro che la differenza tra l'espressione di un dissenso e la capacità di misurarsi con il consenso dei cittadini è il tema che interpella qualunque

altre che si pongono questo interrogativo: come posso io, che non progetto di candidarmi domani alle elezioni su una piattaforma diversa da quella che attualmente non condivido, presentarmi presentarmi davanti alla mia coscienza, alla vita parlamentare e agli elettori con le mie opinioni e un grado decente di rappresentatività e credibilità? Questo mi pare il punto politico che ci viene posto oggi; sarebbe sbagliato sottovalutarlo, colleghi.

voti, per convincimento o piuttosto per convenienza, ovvero che si spostano posizioni dalla maggioranza all'opposizione, o viceversa,

si chiede quanto possa rappresentare i suoi elettori nel momento in cui vive un dissenso politico. Questo è un tema di primaria importanza e, vorrei ringraziare il senatore che respingeremo la sua richiesta di dimissioni e il mio apprezzamento per le motivazioni che egli ha portato, perché sono prova di sensibilità, di onestà politica di civiltà politica, che si aggiungono ovviamente a quei caratteri di qualità professionale, scientifica e parlamentare che tutta l'Aula del Senato mi pare gli riconosca. *(Applausi

prendo davvero solo pochi minuti del vostro tempo per illustrarvi le motivazioni della mia lettera di dimissioni. Nel corso di questa prima parte della legislatura, credo che i colleghi della maggioranza, in particolare quelli della Commissione bilancio, abbiano sperimentato la mia nettezza nel contrastare interventi di politica economica del Governo che ritenevo contrari all'interesse collettivo. In maniera non dissimile, i miei colleghi di partito hanno potuto registrare il mio dissenso rispetto a modalità di essere o di fare opposizione che ritenevo sterili, se non contrarie all'interesse generale. Diversamente che nel primo caso, nel secondo il mio dissenso si è espresso molto raramente in modo pubblico, perché è mia convinzione che la disciplina di Gruppo sia in tempi normali funzionale al corretto funzionamento di questa istituzione. Più in generale, tanto i primi, i colleghi della maggioranza, quanto i secondi, i miei colleghi di partito, hanno avuto più volte la pazienza di sopportare le mie preoccupate considerazioni sulle prospettive del Paese, in un momento che considero veramente di straordinaria delicatezza per il Paese stesso. Mi hanno visto sottolineare, ripetutamente e con forza, la distanza tra le scelte - tanto del Governo quanto dell'opposizione - e le politiche di impronta schiettamente liberale di cui questo Paese da 15 anni, ed ancor più in questo momento, avrebbe estremo bisogno, se possibile nei

come osservano gli storici dell'economia l'Italia, che nella seconda metà del '900 era passata dalla periferia al centro del mondo, ci metterà solo pochi lustri a ritornare dal centro alla periferia. In questo contesto, ai parlamentari si richiederebbe, oltre al rigore personale che certamente li contraddistingue tutti, anche una piena e totale indipendenza di giudizio, in grado di evitare quella che a molti spesso appare, a seconda dei casi, come la miope rigidità o, se volete, la boriosa debolezza dei contrapposti schieramenti, e in grado di evitare che questo si traduca a sua volta, come spesso purtroppo accade, in un danno per la collettività e in un pregiudizio per l'interesse nazionale. Questa indipendenza di giudizio - e qui mi riferisco solo ed esclusivamente a me stesso: non estendo questa argomentazione a nessun altro - trova un limite invalicabile nell'attuale legge elettorale, che priva i parlamentari della legittimità popolare senza la quale, e parlo nuovamente per me, indipendenza di giudizio, con buona pace del dettato costituzionale. Avendo vissuto nel 2001 l'esperienza del collegio uninominale, mi sento oggi - e parlo ancora una volta di me non vedo altro modo per riacquistare anche solo in parte la mia libertà di azione e di giudizio, se non quello di rinunciare alla nomina. Credo di aver espresso con chiarezza, come mi è capitato di fare altre volte, la mia opinione e i miei intendimenti.

rimarrà certamente oggi irrisolto, ma non per questo mancherà di richiedere, in tempi io credo e mi auguro brevi, una soluzione. Ringrazio lei, signor Presidente, e tutti i colleghi per l'attenzione che mi avete dedicato.

I senatori favorevoli ad accogliere le dimissioni premeranno il tasto verde al centro della postazione di voto; i senatori contrari premeranno il tasto rosso a destra; i senatori che intendono astenersi premeranno il tasto bianco a sinistra. Poiché si tratta di una votazione a scrutinio segreto, qualunque sia la scelta di voto effettuata, la luce che si accenderà sarà di colore neutro. Dichiaro aperta la votazione.

a convocarsi fin d'ora al fine di procedere all'accertamento del candidato subentrante al senatore Cuffaro.

Onorevoli colleghi, si sono esauriti gli argomenti previsti dal calendario per la settimana corrente diversi dal sindacato ispettivo.

è stato messo sotto processo per Tangentopoli: ha subito 21 processi ed ha avuto 21 assoluzioni. Finalmente, dopo 15 anni, Nello Polese può tornare alla politica. La sua vita politica è stata strozzata da una serie di processi che si sono rivelati tutti assolutamente sbagliati. Non è questo l'unico caso, ed io avevo già preso la parola a proposito di Rino Formica, che ha aspettato 18 anni prima di essere assolto: quindi, gli hanno rovinato la vita. Naturalmente, voglio citare anche Calogero Mannino, che ha aspettato anche pare, 15 anni per ricevere un'assoluzione. Sono molto contenta, perché ritorna un politico importante, a sostegno di Caldoro. L'uscita dalla politica di Polese, infatti, ha contribuito all'elezione di Bassolino e

terribile, che racconta della violenza del nostro secolo, anche nei Paesi evoluti: spesso è una violenza sugli uomini, altre volte è una violenza sugli animali.

alla fine dell'aprile scorso, perché non più funzionali al divertimento di quanti si erano recati alle Olimpiadi di Vancouver. Quei 100 cani costavano troppo e, in una società evoluta e colta come quella canadese, non c'erano possibilità di adozione o altre soluzioni se non quella dell'uccisione diretta e violenta di queste povere bestie. Credo che nel nostro secolo un'attenzione diversa dovrebbe essere rivolta agli uomini, alle donne e ai bambini, ovviamente, ma anche agli animali d'affezione, quindi che questo disagio si possa raccontare anche con un atto preciso di quest'Assemblea nei confronti del Governo canadese, affinché si proceda con la massima attenzione possibile al rispetto dei diritti degli animali e delle convenzioni internazionali che li tutelano.

del 22 settembre 2010, e si riferisce al finanziamento dei patti territoriali, in generale, e del genovese, in particolare.

si riferisce a un paradiso fiscale, come Santa Lucia. In questo caso il paradiso fiscale è Antigua, dove sappiamo esserci alcuni possedimenti del Presidente del Consiglio,